Nella seduta pomeridiana di oggi, con chiusura alle ore 22 ove necessario, riprenderà l'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge recante sospensione dell'efficacia di disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Se necessario**,** l'esame degli articoli e degli emendamenti proseguirà nella seduta pomeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre, nel corso della quale avranno comunque luogo le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento. A tal fine la seduta di domani potrà eventualmente proseguire fino alle ore 21. La mattinata di domani sarà invece riservata ai lavori delle Commissioni permanenti. La mattinata di domani sarà invece riservata ai lavori delle Commissioni permanenti. Giovedì 5 ottobre, alle ore 10, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni al Senato sulla vicenda Telecom. Potrà poi intervenire un senatore per Gruppo, per non più di 15 minuti (20 minuti complessivi agli oratori del Gruppo misto). Il dibattito, che non prevede votazioni, avverrà con trasmissione diretta televisiva. Nella seduta pomeridiana di martedì 10 ottobre sarà discussa la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, per il cui esame si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nel corso della prossima settimana saranno poi esaminati il decreto-legge sulla detraibilità dell'IVA nonché i disegni di legge e i documenti istitutivi di Commissioni di inchiesta, già previsti dal calendario corrente. Nella giornata di mercoledì 11 ottobre saranno poste all'ordine del giorno le dimissioni reiterate dai senatori Malabarba e Livia Turco. Nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 12 ottobre saranno esaminate le mozioni sulle vicende connesse al discorso tenuto da Papa Benedetto XVI a Ratisbona. Nelle sedute pomeridiane di giovedì 5 e 12 ottobre, il sindacato ispettivo comprenderà anche interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento. Infine, il calendario potrà essere integrato con la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

nella seduta antimeridiana del 28 settembre è proseguitala votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Il relatore ha presentato l'emendamento 1.600 e ha chiesto di intervenire per illustrarlo. Ne ha facoltà. signori del Governo, onorevoli colleghi, oltre ad illustrare rapidamente questo emendamento, fornirò qualche ulteriore notizia sui lavori che in sede informale la Commissione giustizia sta svolgendo, come detto alla fine della precedente seduta. È stata raggiunta un'intesa per quanto riguarda la riforma del decreto legislativo n. 106 del 2006, che è quello che concerne l'organizzazione delle procure. Nel disegno di legge si chiedeva la sospensione anche di questo decreto, insieme agli altri due

che tiene conto dei diversi orientamenti emersi al riguardo. Il punto fondamentale della materia è che per la magistratura non sussiste, già nella stessa Costituzione, la soggezione esclusivamente alla legge.

per evidenti ragioni. Nessuno può dare direttive al giudice nella funzione giudicante sia essa monocratica o collegiale, mentre nell'attività della procura della Repubblica è giusto che ci sia una struttura, un'organizzazione cui possano essere date La formulazione che è stata trovata modifica il decreto n. 106 eliminando un eccesso di gerarchizzazione che in esso era contenuto. Approvando questo emendamento viene meno naturalmente la sospensione del decreto in questione. altresì, signor Presidente, l'accantonamento degli emendamenti che riguardano il decreto n. 109 in materia di procedimento disciplinare. Nel confronto che si è appena concluso, nella sede informale della Commissione giustizia, si sono verificati testi e soluzioni che rendono non sicura, ma possibile un'intesa su questo punto. Quindi, signor Presidente, se lei e l'Aula siete d'accordo, proporrei l'accantonamento degli emendamenti che si riferiscono esclusivamente al decreto n. in modo che nella seduta pomeridiana prevista per domani saremo in grado di dire se anche su questo decreto si è raggiunta l'intesa ovvero no. Infine, signor Presidente, preannuncio fin d'ora il mio parere favorevole agli emendamenti soppressivi dell'articolo 3

positivo in questo campo e contribuirebbe anche a un più sollecito esame del provvedimento. Ringrazio tutti per la precisa attenzione che è stata concessa a queste mie considerazioni.

il residuo di una campagna elettorale consumata da poco, ma che è anche il retaggio di una contrapposizione - che è stata violentissima nella scorsa legislatura - su una materia come questa, che tocca direttamente i cittadini. Presidente, niente più del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, riguarda direttamente i cittadini, compresi i colleghi Izzo e Pisanu, che invece non sono molto interessati e continuano a chiacchierare alle mie spalle. Tale

stato possibile perché c'è stata una grande disponibilità dell'Aula a recepire un'esigenza, c'è stata una grande disponibilità da parte del relatore a favorire una sintesi c'è stata una grande disponibilità di tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione ad impegnarsi concretamente sul terreno di una normativa assolutamente modificata per determinare quelle condizioni che i cittadini, in qualche modo, ci chiedevano. È chiaro che molto ha fatto anche la Presidenza del Senato, che in ogni modo, con la sua assoluta discrezione e con la sua capacità di non essere assolutamente mai giocatore in campo, ma con una serie di indicazioni tacite, ha favorito un approccio di questo tipo. Un altro ringraziamento sicuramente è dovuto al ministro della giustizia Clemente Mastella che ha voluto che questo metodo fosse perseguito: metodo che poi, signor Presidente, era stato invocato

di creare un'uniformità di gestione delle procure. Ciò significa immaginare che le indagini vengano gestite tutte allo stesso modo

compartecipazione nella gestione delle procure, per non accentrare esclusivamente nelle mani del procuratore capo un potere che invece volevamo fosse

il sostituto procuratore, possa nascere un rapporto più fecondo, proficuo e corretto. L'unica logica che ha ispirato queste misure è quella del cittadino. Sono convinto che il grande sforzo che il Senato ha messo in campo rispetto a questo provvedimento

quindi soddisfatto dell'iniziativa che è stata portata avanti e sono convinto che alla lunga anche coloro che adesso sono dubbiosi comprenderanno che questa è un'iniziativa che ha la capacità di far materializzare la politica buona, che dovrebbe essere sempre capace di privilegiare le scelte

sia perché testimonia la possibilità di intesa su problemi fondamentali, qual è quello dell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, sia perché fa giustizia di tanti estremismi che possono trovare posto nella campagna elettorale, ma che non devono trovare posto nelle Aule del Parlamento, nelle concezioni contrapposte, spesso frutto di ideologia e di posizioni eterodirette. Esprimo soddisfazione perché ho sentito della condivisione della necessità di una uniformità d'indirizzo nell'esercizio dell'azione penale da parte di un ufficio così fondamentale come la procura della Repubblica. Repubblica. Esprimo soddisfazione perché, in definitiva, l'impianto complessivo rimane assolutamente identico nella sostanza e quindi viene ad essere riconosciuta la bontà di quell'impianto in un primo tempo assolutamente demonizzata. Così non è nella realtà dei fatti perché non si è verificato alcun problema negli uffici di procura: non abbiamo notizie di rivolte di pubblici ministeri, di incidenti di percorso. Alcuni procuratori, anzi,

il procuratore della Repubblica continua a rimanere titolare esclusivo dell'azione penale (ciò dà senso all'uniformità di indirizzo alla base di questo decreto delegato) il magistrato, invece che delegatario, diventa assegnatario. Insomma, a ben vedere si tratta soltanto di una differenza nell'uso della terminologia. Potremmo anche discettare sulla sostanziale diversità tra i due termini, ma in realtà ci si deve attenere a quei criteri indicati dal procuratore della Repubblica che potrà, anche in questa occasione con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione. la sintesi raggiunta permette di far sì che non vi sia nessun ricorso ad alcuna autorità, sia essa il procuratore generale della Cassazione (come nel testo vigente), sia esso il Consiglio superiore della magistratura o eventuali altri. Questo significa rafforzare la figura del procuratore della Repubblica senza con ciò far venire meno le possibilità già previste oggi dall'ordinamento, quali: un'eventuale denuncia penale

probabilmente, non saremmo stati così costretti dalla presenza del provvedimento in Aula. Avremmo potuto ragionare con maggiore tranquillità e magari avremmo potuto pensare anche all'impianto complessivo. Rimane, comunque, l'ottimo risultato di questo accordo; rimane una nuova visione degli uffici della procura che evita anche quei protagonismi, quella ricerca di visibilità mediatica attraverso un unico portavoce, sia esso il procuratore della Repubblica o un suo delegato. Esprimo, infine, soddisfazione perché in questo modo viene ad essere confermato l'impianto della riforma proposta dall'allora ministro della giustizia Castelli e dalla Casa delle Libertà.

non lo riteniamo motivo per il quale si debba andare oltre il profondo rammarico per quanto è accaduto. Lo faccio perché ho l'impressione

non c'è volontà di protagonismo, di partito o di Gruppo parlamentare, in ordine a ciò che sta avvenendo in riferimento alle procure della Repubblica.

che fosse possibile trovare un'intesa di largo consenso parlamentare su provvedimenti istituzionali come quello relativo all'ordinamento giudiziario. Siamo quindi particolarmente lieti per aver concorso, in modo forse determinante, a tale risultato. Il ministro Mastella ricorderà

Siamo quindi particolarmente lieti che quel supplemento abbia prodotto un risultato utile ed è la ragione per la quale, nel rivendicare in parte il merito di questo risultato molto importante, esprimo l'auspicio che anche per ciò che concerne l'azione disciplinare

Voglio garantire che il Gruppo UDC continuerà in queste ore e domani mattina a ricercare un'intesa dignitosa, sapendo che questa richiede necessariamente che le due parti si ritrovino su un punto d'accordo al quale nessuna delle due sarebbe stata da sola desiderosa

Se così non dovesse essere, do però per scontato che faremo di tutto perché anche su questo argomento si possa trovare un punto di equilibrio. Ancora una volta questo equilibrio istituzionale, avvenendo nel pieno di uno scontro politico molto forte sulla finanziaria presentata dal Governo, dimostra che ci si può attenere ad una distinzione tra gli aspetti istituzionali, per i quali è necessaria costituzionalmente un'intesa

ha colto un punto: in Aula non è stato commemorato e ricordato l'alpino Vincenzo Cardella. Ieri mattina, a nome del Senato, ho portato la nostra solidarietà ai familiari ed ho visitato la camera ardente.

Signor Presidente, la prima delle proposizioni contenute nel disegno di legge proposto dal guardasigilli, il ministro Mastella, era volta a sospendere l'efficacia del decreto delegato con cui, in attuazione della cosiddetta riforma Castelli dell'ordinamento giudiziario, veniva disegnato un nuovo modello dell'ufficio del pubblico ministero centrato sul principio che titolare esclusivo dell'azione penale è il procuratore della Repubblica, che quindi incarna l'ufficio stesso. La proposizione del disegno di legge era dunque quella di sospendere l'efficacia di questo complesso normativo e segnatamente degli otto articoli di cui lo stesso è composto. Il risultato a cui perveniamo, attraverso quella che confido essere l'approvazione dell'emendamento 1.600, firmato dal relatore in attuazione di un accordo ampio intervenuto tra le forze politiche, tra le forze politiche, è quello del mantenimento, così come sono, degli articoli da 2 a 8 del decreto delegato di cui sto parlando, e quindi, del mantenimento così come dell'intero modello dell'ufficio del pubblico ministero come disegnato dalla maggioranza e dal Governo di centro-destra nella passata legislatura, con riferimento ad un ufficio centrale nel sistema di funzionamento della nostra giustizia. Con la modifica del primo articolo di questo decreto delegato si interviene in relazione a tre punti precisi. Il primo è la soppressione delle parole «sotto la propria responsabilità»; il procuratore della Repubblica resta titolare esclusivo di un'azione penale resta titolare esclusivo di un'azione penale che non esercita più solo sotto la propria esclusiva responsabilità, ma sotto la responsabilità condivisa sua e di coloro i quali sono parte del suo ufficio. La seconda modifica introdotta riguarda una correzione puramente lessicale. Il sottosegretario Scotti ha sottolineato l'ipertrofia legislativa che era contenuta nelle parole «nei modi e nei termini stabiliti dalla legge»; abbiamo quindi rimosso queste parole. La terza modifica è quella che forse ha un significato più incisivo, nel senso che stabilisce che i contrasti all'interno delle procure della Repubblica, se sono contrasti che rimangono nell'ambito della fisiologia dialettica, si risolvono con la decisione del titolare esclusivo dell'azione penale, cioè del procuratore della Repubblica. Se invece è una dialettica che trascende la fisiologia e precipita nelle patologie, allora saranno risolti attraverso i sistemi che il sistema - le chiedo scusa per il bisticcio, signor Presidente - prevede per questi casi: il ricorso al procedimento penale e il ricorso al procedimento disciplinare. Come si vede, abbiamo una larghissima parte dello strumento normativo che avevamo proposto che rimane inalterata e la parte che viene modificata lo è in in termini migliorativi, per quanto ci sembra, in alcuni aspetti e in termini marginali per altri. Il tutto attraverso una proposta puntuale che abbiamo presentato proprio noi, senatori di Alleanza Nazionale. Credo che il Gruppo di AN possa ascriversi un po' la primogenitura

parola agli atti. Credo che da parte di chi mi ha preceduto sia stata esternata una giusta e corretta soddisfazione per essere arrivati ad un fatto positivo, come è stato ricordato, *in* *primis* per i cittadini, ma - credo - anche per il buon funzionamento degli uffici della procura. Se possibile, per me la soddisfazione è doppia,

erano, evidentemente, strumentali e false. Si potrebbe aprire una pagina polemica, ma non credo sia il caso, visto che guasterebbe la nuova atmosfera di positività che si è aperta sul provvedimento. Credo che sia questo l'aspetto che va colto e i i sassolini nella scarpa ce li toglieremo in un secondo tempo, in sedi magari più appropriate. Dunque, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.600

ma che è nato da un incontro e da una concordanza non semplice tra maggioranza e opposizione. Tale intesa riguarda l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e ruota intorno ad una visione unitaria dell'attività requirente e dell'assetto delle procure. Il procedimento viene assegnato dal procuratore della Repubblica al suo sostituto. Il procuratore della Repubblica definisce i criteri per l'esercizio dell'azione penale da parte di ciascun magistrato del suo ufficio; egli ha anche un potere di revoca del procedimento ed è data la possibilità al sostituto di rivolgere proprio al procuratore della Repubblica doglianze ed osservazioni ove egli ritenga non giusto l'esercizio del potere di revoca. É evidente che, in caso di contrasto sulla base dei principi fissati dell'ordinamento, chi decide, chi dirime il contrasto è l'organo di governo autonomo della magistratura. Per queste ragioni abbiamo ritenuto che l'intesa raggiunta fosse ragionevole e, sempre per queste ragioni, stiamo prendendo un po' di tempo, all'inizio di questa seduta, per portare in Aula la scelta che si è compiuta, le ragioni che ci hanno indotto alla convergenza ed anche la valutazione di ciascuna forza politica su questo testo. Naturalmente, rimane tra noi e il centro-destra, su questo tema specifico ma più in generale sulla tematica dell'ordinamento giudiziario, una vasta area dissensi; permangono opinioni alternative, una visione dei problemi della giustizia che ci allontana dalle posizioni espresse dal centro-destra e che allontana il centro-destra dalle nostre

le premesse culturali proprie della nostra e della vostra coalizione in ordine ai problemi della giustizia ma, tenendo conto di queste differenze, è ancora più rilevante, mi sembra, il lavoro comune che stiamo cercando di condurre. Naturalmente, per chiarezza, abbiamo rinviato a domani mattina la discussione su alcuni aspetti relativi alle norme in materia disciplinare, perché questa materia è più complessa e perché in tale campo è più difficile superare le divergenze; ma noi confidiamo sulla possibilità che le divergenze siano superate perché anche su questo tema si ravvisi un punto di incontro. Su questo intendimento, che naturalmente non significa in alcun modo offuscare le differenze e le peculiarità delle nostre rispettive concezioni, vorrei rassicurare anche il collega Manzione. Fin dall'inizio vi è stata la nostra disponibilità alla convergenza, naturalmente tenendo fermi i principi dai quali muoviamo,

ascoltato prima il senatore Salvi e poi il senatore Brutti affermare che tra il centro-sinistra e il centro-destra vi è una diversa concezione del mondo della giustizia. Questo è sicuramente vero perché, senza voler fare alcuna polemica, non da entrambe le parti si immagina il mondo della giustizia in assoluta libertà o in assoluta assenza di correlazioni con interessi di parte. n. 160, ministro Mastella, è quello che riguarda più da presso la vita e la carriera dei magistrati e costituisce il cuore della riforma dell'ordinamento giudiziario. Fra poco voteremo e, se la maggioranza avrà i voti, questo decreto legislativo verrà sospeso. Vede, ministro Mastella, seguendo sempre il suo intervento, mi consenta di dirlo, da politico intelligente, ci sono dei nodi che devono essere sciolti e che lei si è ben guardato dal chiarire. È strano, ministro Mastella: lei afferma di condividere l'impianto previsto nel decreto legislativo per l'entrata in magistratura e cioè, sostanzialmente, di immaginarlo come un concorso di secondo grado. L'unica eccezione e l'unica difformità rispetto al testo della riforma Castelli è quello che - devo dire con non eccessiva bontà - il senatore Salvi ha inteso definire una *boutade*: cioè consentire a chi è consigliere comunale, provinciale, regionale o deputato di entrare in magistratura, mi auguro, evidentemente, avendo sempre, almeno, la laurea in giurisprudenza. tanto di una *boutade*, se è vero che questo è un requisito richiesto, ad esempio, per l'entrata nella giustizia amministrativa. Di sicuro, però, ministro Mastella, lei dimentica che nella precedente legislatura all'unanimità la Camera dei deputati - solo la Camera, ahimè! - ha approvato una proposta di legge tutta tesa ad impedire qualsiasi forma di commistione tra la politica e i magistrati.

Tuttavia, sostanzia questa separazione dando la possibilità ogni tre anni ad un magistrato di passare dall'ufficio del pubblico ministero all'ufficio del giudice e, conseguentemente, di ritornare a fare il pubblico ministero con l'unico limite del cambiamento di distretto. Credo che i suoi uffici l'abbiano informata del fatto che il cambio da un ufficio all'altro avviene solo nei primi anni della carriera ed è strettamente funzionale al posizionamento in un posto «più vicino a casa», o ha luogo per motivi di carriera. Spesso abbiamo visto procuratori della Repubblica diventare presidenti del tribunale o consiglieri istruttori divenire procuratori della Repubblica nello stesso identico circondario, evidentemente con buona pace di quel concetto reale o di apparenza che è la terzietà del giudice prevista dall'articolo 111 della Costituzione. Allora, ministro Mastella, ci spieghi - perché quanto meno gli avvocati sono interessati a saperlo che tipo di separazione di funzioni lei immagina: se si tratta, cioè, di una separazione, per così dire, trotterellante da un distretto all'altro, ma che vede il giudice e il pubblico ministero sostanzialmente identici a come erano prima della riforma Castelli, o qualcosa di diverso. Tenga presente, ministro Mastella, che quando si è immaginata la separazione delle funzioni, peraltro in ossequio a una chiara sentenza della Corte costituzionale,

che il sistema concorsuale è tale da impedire ai magistrati di dedicare il loro tempo all'attività lavorativa. Non è vero, non è assolutamente vero. Il sistema concorsuale previsto dalla legge è esattamente quello disegnato da un autorevole esponente di Magistratura democratica, il consigliere Nello Rossi, ed è esattamente quello auspicato dal presidente Marvulli, cioè che vi sia una commissione filtro che possa valutare compiutamente l'attività realmente svolta sul campo dai magistrati, così da poter proporre al Consiglio superiore della magistratura una terna all'interno della quale il Consiglio stesso possa adottare le sue scelte. scelte. Ministro Mastella, per troppi, troppi, troppi anni il Consiglio superiore della magistratura è stato la fonte del maggiore inquinamento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, perché troppi, troppi, troppi, davvero troppi sono i casi in cui magistrati di assoluto valore non hanno avuto soddisfazione alle proprie aspirazioni perché erano fuori delle logiche correntizie o non frequentavano salotti politici.

di fare il consigliere istruttore di Palermo, successivamente quella a fare il procuratore nazionale antimafia e, principalmente, trovandosi sottoposto ad una procedura di trasferimento d'ufficio solo perché si era reso responsabile di imputare di calunnia tale Pellegriti invece di imputare per associazione mafiosa il senatore Andreotti.

perpetuare dando sfogo alle logiche di potere della corrente, ma principalmente esaltando il ruolo di compressione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che si gioca tutto all'interno del Consiglio superiore.

ma dovrebbe ricordare che il Presidente della Repubblica, nel messaggio di rinvio alle Camere, puntò la sua attenzione proprio su quell'ufficio, considerandolo in contrasto con la Costituzione perché compressivo dell'autonomia

Di fronte a me c'è un voto espresso da qualche entità non materiale. Vi prego di togliere la scheda.

Presidente, mi scusi, ma è veramente disdicevole che noi si debba far polemiche in quest'Aula sui doppi voti.

Signor Presidente, signor Ministro, vorrei attirare l'attenzione del Governo e dei colleghi della maggioranza sulla circostanza che il Capo II del decreto delegato contiene esclusivamente un'elencazione di funzioni secondo i paradigmi già oggi esistenti. Infatti, quando si che le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni, di magistrato di sorveglianza si fotografa esattamente la situazione attuale stesso vale per le funzioni requirenti di primo grado e per le funzioni giudicanti di secondo grado, e così via. È un capo assolutamente ininfluente e, come suole dirsi, neutro, che definisce esclusivamente le funzioni secondo quanto già esiste oggi. Allora, mi chiedo qual è la necessità di questa sospensione quando poi dovrà certamente essere riproposta perché non si potrà diversamente, al di là delle opinioni diverse sulla separazione o distinzione delle funzioni, sulla loro reversibilità o meno, sul modo di accedere alla magistratura.

in carriera, anche remunerativa, dei magistrati. Mi pare, da quanto ho letto, che vi siano anche degli interventi proprio per quanto riguarda le varie funzioni. questo voto sarebbe importante perché invece statuirebbe la volontà del Parlamento in tal senso. Quindi, inviterei il relatore e il Governo a meditare sulla questione. Tra l'altro, *in cauda venenum*, dico che il cattivissimo ministro Castelli e la Casa delle Libertà si erano ben guardati dal toccare gli stipendi dei magistrati, i quali adesso hanno appoggiato in maniera eclatante il Governo di sinistra che li ripaga con questo premio e taglia loro gli stipendi. Bene, credo

Signor Presidente, questo emendamento punta ad attuare concretamente quella meritocrazia e quella possibilità di selezione, e quindi di premio, della della quale si parla tanto ma di cui pochi tendono all'attuazione. Ci dobbiamo intendere e chiarire: oggi i concorsi per titoli sono quelli che consentono di arrivare in appello e in Cassazione soltanto attraverso l'anzianità e la mancanza di demerito,

Gli unici due concorsi in più introdotti dalla riforma Castelli sono quelli che riguardano la possibilità di arrivare alle funzioni di giudice d'appello e di legittimità prima del tempo consentito. Facciamo venir meno quella gerontocrazia che impera anche in magistratura e che fa arrivare, evidentemente, in Cassazione ad un livello di età e di carriera in cui non sempre si riesce a mantenere intatto quello spirito e quella capacità che ogni magistrato dovrebbe continuare ad avere in ogni momento della sua carriera.

in Cassazione o se non è più utile farlo arrivare prima alla Corte di cassazione per dare maggior lustro all'organo e dare più forza, slancio e incisività alla giurisprudenza della Cassazione. questo ci dobbiamo interrogare: certamente questi concorsi - che comportano, a differenza degli altri, anche degli esami, perché comunque permettono un'anticipazione di carriera - servono a selezionare magistrati per dei livelli di straordinaria importanza, quali sono l'appello e le funzioni di legittimità. Non servono certamente a far fuggire dalle funzioni di primo grado, che sono anch'esse di straordinaria importanza, come molti colleghi hanno sostenuto,

di cui tanto parla l'Associazione nazionale magistrati, ma solo in termini generali e di cui tanto parlano tutte le forze politiche, ma che in quest'occasione viene attuata concretamente.

da cui sono stati originati i decreti delegati che hanno attuato la cosiddetta riforma Castelli, si fa carico di introdurre nell'ordinamento delle disposizioni che consentano al legislatore, o per meglio dire al legislatore delegato (cioè al Governo), di intervenire per stabilire la disciplina transitoria eventualmente necessaria per traghettare le vecchie norme dell'ordinamento vigente alle nuove norme dell'ordinamento riformato, oltre che per introdurre le eventuali disposizioni di coordinamento ed

dopo che fosse entrato in vigore l'ultimo dei vari decreti delegati previsti per l'attuazione della riforma. Il Governo, con il disegno di legge ora proposto dal Ministro guardasigilli, ha prorogato questo termine con la stessa logica di proroga e la stessa logica di sospensione.

sia prevista la possibilità per il Governo di intervenire con specifiche norme transitorie di coordinamento ed abrogative non nel termine di un anno e novanta giorni

ma in un termine contenuto dal momento in cui ciascun decreto delegato acquista efficacia, perché è in quel momento che si concretizza la necessità di una disciplina transitoria che operi - come ho detto - da traghetto fra il vecchio e il nuovo ordinamento.

Presidente, si tratta di una questione meramente tecnica in merito alla quale pregherei il relatore e il Ministro di ascoltarmi un attimo. Questa è sostanzialmente una norma di chiusura, perché noi siamo intervenuti in maniera assolutamente complessa e quindi è evidente che durante i lavori in Aula non è possibile valutare tutte le ricadute che questi decreti e questa riforma possono avere. Viene quindi giustamente delegato il Governo affinché possa intervenire il più rapidamente possibile con norme di coordinamento, perché sicuramente si potranno rilevare delle discrepanze. giorni era un termine che sembrava a metà strada tra la necessità di agire urgentissimamente e invece la necessità del Governo di poter valutare e poi intervenire in maniera meditata sulla materia. Credo che sei mesi sia invece un termine che procrastina troppo il regime transitorio; rischieremmo di avere per sei mesi delle norme che non sono coordinate tra loro. Per tale ragione pregherei veramente il relatore e il Governo di ripensarci e di mantenere il termine di novanta giorni. Non c'è assolutamente nulla di politico in tutto ciò, è soltanto una questione di natura tecnica.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti del senatore Formisano.

la sorte che ha avuto, dal punto di vista della proponibilità o dell'improponibilità, l'emendamento 4.0.600 del Governo. è stato dichiarato proponibile. stretti criteri di pertinenza dettati dal nostro Regolamento, con cui lei ha inteso interpretare tutti gli emendamenti che intervenivano in maniera assonante a questo.

il documento corretto; poi vedo l'annesso III e anche qui non vi sono interventi modificativi. Non Non credo di avere documenti non aggiornati. Non mi sembra che vi sia stata nessuna modifica in corso d'opera. Mi sembra semplicemente che si tratti di un argomento aggiuntivo - il Governo ha presentato giustamente un emendamento aggiuntivo - che avrebbe dovuto

fatto sviluppare poi i lavori, tutti gli emendamenti che entravano nel merito erano stati dichiarati improponibili, così è stato fatto nell'altra seduta; mentre questo, poiché riguardava soltanto la fissazione dei termini, accettato e quindi lo abbiamo mantenuto per la votazione. Questa è stata la ragione, senatore Caruso, di una decisione già presa.

POSSA *(FI)*. Signor Presidente, noto con piacere che sono presenti in Aula una dozzina di illustri rappresentanti del Governo. Credo che non si sia mai verificata nella scorsa legislatura una simile presenza in massa di membri del Governo.

elettronico, dell'articolo 4. Dichiaro aperta la votazione.

che un aereo turco, con due dirottatori a bordo, è atterrato a Brindisi, l'aeroporto è stato chiuso, il veicolo è stato circondato.

La seduta è ripresa. Comunico all'Assemblea che ho avuto contatti diretti con il Ministro dell'interno